nel quadro della forte azione a difesa delle libertà fondamentali a livello internazionale, il Ministero degli affari esteri segue con grande attenzione la vicenda che ha visto coinvolta Maryam Bahrman, figura importante della lotta per la promozione dei diritti umani ed in particolare contro la discriminazione femminile in Iran. Come ricordato dagli onorevoli interroganti, la signora Bahrman si è, infatti, distinta come segretario generale dell'Organizzazione per la parità delle donne, chiusa su intervento delle autorità iraniane nel 2007, e come promotrice della campagna «Un milione di firme per l'uguaglianza», condotta allo scopo di sensibilizzare il Governo di Teheran al pieno rispetto delle convenzioni sui diritti umani ratificati dall'Iran. Nell'ambito della sua attività per la tutela delle libertà fondamentali si iscrive anche la partecipazione, nel marzo del 2011, della signora Bahrman a un ciclo di conferenze organizzato a New York dalla Commissione sulla condizione delle donne delle Nazioni Unite. In tale contesto ella ha preso parte anche ad un seminario organizzato da AIDOS (Associazione italiana donne per lo sviluppo) con un apprezzato intervento sulle discriminazioni contro le donne le donne nell'accesso alle nuove tecnologie informatiche, ribadendo l'auspicio di una revisione delle severe leggi islamiche sulla condizione femminile vigenti in Iran e invocando pari diritti per le donne, sia nel mondo del lavoro che della società in generale. Ha quindi destato grande perplessità e apprensione l'arresto della signora Bahrman l'11 maggio 2011 da parte delle forze dell'ordine iraniane che, prelevandola dal suo domicilio a Shiraz, l'hanno trasferita presso un centro di detenzione della medesima città, dove si trova tuttora reclusa, con l'accusa di aver commesso non meglio precisati atti contro la sicurezza nazionale. Oltre che al suo impegno in favore dei diritti delle donne e alla sua partecipazione alle conferenze della Commissione ONU, l'arresto potrebbe essere collegato alla lettera che, pochi giorni prima, la signora Bahrman aveva indirizzato - pubblicandola anche sul suo *blog* personale - al leader dell'Onda Verde Mousavi e a sua moglie Rahnavard. Nella lettera pubblica, l'attivista esprimeva loro solidarietà, contestando gli arresti domiciliari loro imposti dal febbraio 2011 e auspicando che «questi giorni amari possano essere presto dimenticati». La Farnesina si è subito attivata, attraverso la nostra ambasciata in Iran, coinvolgendo i partner comunitari per un'azione corale dell'Unione europea nei confronti delle autorità iraniane. Su iniziativa della nostra rappresentanza, il caso della signora Bahrman è stato inserito tra quelli più attentamente monitorati dalle ambasciate europee a Teheran. I capi missione UE ne hanno discusso anche recentemente registrando unanime apprensione per l'assenza di aggiornamenti sullo stato della donna e per l'incertezza su tempi e modalità di un eventuale processo a suo carico. Sempre grazie al contributo dell'Italia, l'Alto rappresentante UE Ashton, in una dichiarazione del 6 luglio scorso, ha invocato il rilascio della signora Bahrman insieme ad altre quattro donne iraniane colpite negli ultimi mesi da una recrudescenza della repressione iraniana contro il mondo intellettuale femminile. In questo quadro, la Farnesina rimane impegnata a seguire la vicenda in stretto raccordo con i partner comunitari, tenuto conto che le autorità iraniane hanno in passato dimostrato di tenere in considerazione il danno di immagine derivante da circostanziate denunce a livello internazionale. Questa azione si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative sostenute dal Governo italiano, in particolare a livello comunitario e nell'ambito dei competenti organismi delle Nazioni Unite, per promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Iran. La situazione complessiva nel Paese continua, infatti, a suscitare forte preoccupazione. La repressione degli oppositori politici si è intensificata a seguito delle elezioni presidenziali del giugno 2009. Numerosi esponenti sono tuttora in carcere, spesso in gravi condizioni detentive. La decisione del leader supremo Khamenei dello scorso 27 agosto di liberare un numero non ben definito (comunque inferiore ai 100) di detenuti politici - inclusi alcuni dissidenti coinvolti nelle proteste che hanno fatto seguito alla contestata rielezione di Ahmadinejad - in occasione del termine del periodo di Ramadan non ha infatti portato ad un miglioramento concreto della situazione. Non è pertanto escluso che il gesto del leader sia da porre nel più ampio quadro dei recenti tentativi del campo conservatore di corteggiare il sostegno, se non di tutti, almeno della parte più moderata dei riformisti, in vista delle prossime elezioni parlamentari di primavera. La cronaca dei giornali internazionali ha registrato, anche in questi mesi, arresti di studenti, avvocati difensori, attivisti dei diritti umani. La maggior parte dei *media* non allineati al regime è stata chiusa, così come gli uffici dei principali partiti politici riformisti. Le statistiche dimostrano purtroppo un incremento delle condanne capitali, spesso per reati connessi al traffico di stupefacenti e a seguito di accusa di insurrezione contro lo Stato. Tra le più recenti iniziative adottate con il contributo italiano, vorrei ricordare la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 12 aprile 2011 con cui sono state adottate misure restrittive (divieto di ingresso e congelamento di eventuali beni posseduti nell'Unione europea) nei confronti di 32 esponenti del regime, ritenuti responsabili di gravi violazioni dei diritti civili. A novembre 2010 l'Italia ha sostenuto l'approvazione, da parte della Terza Commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, della risoluzione di condanna nei confronti dell'Iran, che viene riproposta ogni anno dal Canada e co-sponsorizzata da tutti i Paesi UE. Quest'anno si è ottenuto un consenso crescente (80 voti a favore, 44 contrari e 57 astenuti, a dimostrazione che esiste ormai un'ampia consapevolezza della gravità della situazione. Vorrei anche sottolineare l'accettazione da parte iraniana di 23 raccomandazioni nel corso dell'Esame periodico universale sulla situazione dei diritti umani tenutosi a Ginevra, presso il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, il 15 febbraio 2010. Due di esse sono state formulate su iniziativa dell'Italia per sollecitare la ratifica della Convenzione contro la tortura e sul bando delle esecuzioni di minori, in accordo con l'articolo 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Anche per effetto della pressione esercitata dall' Unione europea, si è ottenuto il significativo ritiro della candidatura iraniana al Consiglio diritti umani per il mandato 2010-2013 e la mancata elezione di un rappresentante di Teheran nella Commissione ONU sulla condizione femminile. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha anche approvato, lo scorso 24 marzo, la nomina di un relatore speciale incaricato di verificare la situazione dei diritti umani in Iran. Da parte italiana si condivide l'opinione prevalente tra i Paesi comunitari, secondo cui denunce e misure sanzionatorie non devono essere fini a se stesse, bensì indurre le autorità iraniane a impegnarsi per migliorare le condizioni dei diritti umani e ad aprirsi al dialogo con la comunità internazionale. Siamo pertanto favorevoli anche a misure parallele - quali seminari di taglio accademico, riunioni a livello esperti dentro e fuori l'Iran, contatti diplomatici regolari - volte a costituire canali di comunicazione attraverso i quali rappresentare le nostre preoccupazioni per i casi di violazione più urgenti ed eclatanti e salvare così vite umane. Occorre infatti evitare un innalzamento del livello di tensione che ponga l'Iran a rischio di rimanere privo di sbocchi politici. In questo senso, l'approccio dell'Italia è fermo nella difesa dei principi tempo, aperto al dialogo per svolgere pressione ed esercitare contestualmente opera di persuasione, in conformità con la tradizionale posizione dell'Italia

disponibile a rispondere alle due interrogazioni, anche se, soprattutto per la concitata situazione che abbiamo vissuto in quest'ultimo periodo,

Certamente, possiamo prendere atto dell'impegno del nostro Ministero degli affari esteri. Tuttavia, penso di dover fare due considerazioni: la prima, a sostegno dell'iniziativa del nostro Paese e della necessità di continuare a sviluppare e incalzare le autorità di

ha avuto la possibilità di accedere alle organizzazioni internazionali. Proprio per questo motivo viene attaccata per attentato terroristico nei confronti dello Stato iraniano e viene anche messo in discussione il ruolo e la funzione di un'organizzazione non governativa come AIDOS. Tutto

della legge sulle organizzazioni non governative, e i servizi segreti stanno cercando di entrare dentro a questa parte

auspicato e formulato per aiutare la crescita della sensibilizzazione della società iraniana, può avere questo ruolo e svolgere questo compito nella propria realtà, ma anche fornire a noi tutti gli elementi di conoscenza per un'azione più efficace.

Signora Presidente, in premessa vorrei ricordare che, allo stato attuale, non è possibile fornire cifre sulla quota di PIL da destinare nel 2015 agli aiuti pubblici allo sviluppo. Come è noto, infatti, la legge di stabilità attualmente in vigore, che di regola ha valenza triennale, si riferisce al periodo 2011-2013, mentre la legge di stabilità per il triennio 2012-2014 è in corso di elaborazione e verrà esaminata dal Parlamento nel prossimo autunno. Vorrei comunque rassicurare l'Aula circa lo sforzo del Governo a mantenere, compatibilmente con le imprescindibili esigenze di risanamento di bilancio dello Stato, gli impegni assunti in materia di cooperazione allo sviluppo. Ne è testimonianza il nostro impegno in materiali salute materno-infantile. Il rapporto diffuso al Vertice di Deauville del luglio scorso sullo stato d'attuazione degli impegni G8 in materia di sicurezza alimentare e salute, rende noto che l'ammontare addizionale per il quinquennio 2011-2015 versato dall'Italia per l'iniziativa in materia di salute materno-infantile adottata al Vertice di Muskoka, è di 75 milioni di dollari. Sempre il Rapporto di Deauville rileva che l'Italia ha erogato, nel biennio 2009-2010, 349 milioni di dollari per 1'«*Aquila Food Security Initiative*» Si tratta di circa l'82 per cento dell'impegno complessivo preso all'Aquila dal Governo italiano, pari a 428 milioni di dollari nel triennio 2009-2011. In ambito G8, l'Italia è il Paese che, assieme al Canada, registra il più alto tasso di esecuzione dell'iniziativa e, tenuto conto delle attività che sono in corso di realizzazione nel 2011, riteniamo di poter portare a compimento gli impegni presi. L'iniziativa dell'Aquila, che è stata lanciata proprio sotto la Presidenza italiana del G8, ha avuto il grande merito di rimettere la questione della sicurezza alimentare al centro dell'agenda internazionale, individuando i principi fondamentali in tema di sviluppo agricolo e sicurezza alimentare, che sono poi stati adottati al Vertice FAO del novembre 2009. L'iniziativa dell'Aquila figura peraltro fra le priorità anche della Presidenza USA del G8 del 2012. Vorrei anche sottolineare come l'Italia, in qualità in qualità di membro dell'Unione europea, ha onorato *pro quota* il proprio impegno contratto con la Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare. Tale impegno, che si sostanzia in un contributo complessivo di 162,3 milioni di euro per il periodo compreso tra il giugno 1999 e il gennaio 2004, pari ad un valore annuo di 36,2 milioni di euro, ha consentito di fornire assistenza alimentare alle fasce più vulnerabili di oltre 80 Paesi in via di sviluppo. Nel periodo compreso tra il gennaio 2004 ed il giugno 2011 non è stato possibile corrispondere le quote per sostenere le attività della Convenzione di Londra, comportando un mancato finanziamento pari a complessivi 271,5 milioni di euro. Le ragioni sono note. Il primo triennio di partecipazione alla Convenzione (1999-2001) è stato finanziato con legge 29

Al termine del primo triennio la Convenzione è stata prorogata con cadenza annuale; si è quindi reso necessario, da parte italiana, provvedere annualmente ad assicurare per legge i relativi finanziamenti. La prima proroga, dal giugno 2002 al giugno 2003, è stata finanziata con la legge 17 giugno 2004, n. 155, per un totale di 36,2 milioni di euro. La seconda proroga, dal giugno 2003 al giugno 2004, è stata in parte finanziata con la legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha previsto degli stanziamenti per 18,1 milioni di dollari. In entrambi i casi veniva statuito che «all'onere derivante dall'applicazione dell'impegno si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario relativo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri». Per mettersi in regola con gli impegni previsti dalla Convenzione l'Italia dovrebbe versare oggi un totale di 271,5 milioni di euro. L'esiguità delle risorse disponibili presso il Fondo speciale di tabella A del Ministero degli affari esteri, nonché le necessità di rigore di bilancio, non hanno consentito negli ultimi anni la presentazione di un provvedimento sulla materia da parte del Ministero degli affari esteri; né sarebbe concepibile, data l'entità delle cifre in gioco, sopperire al mancato finanziamento con i fondi ordinari della cooperazione. Nonostante la difficile congiuntura economica internazionale, l'impegno della nostra cooperazione allo sviluppo per la riduzione dell'insicurezza alimentare e la riduzione della fame nel mondo resta comunque assolutamente prioritario. Per quanto riguarda il Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria, vorrei ricordare come anche questo sia nato nel 2001 proprio su impulso della Presidenza italiana del G8. Il Fondo ha caratterizzato l'azione del nostro Paese in materia di cooperazione allo sviluppo in campo sanitario negli ultimi anni. Tra il 2001 e il 2008 l'Italia ha erogato al Fondo una somma pari a 790 milioni di euro, risultando il terzo principale donatore dopo Stati Uniti e Francia. Il versamento delle quote relative al 2009 e al 2010 è stato anch'esso ostacolato dalle note, pressanti esigenze di risanamento della finanza pubblica, recentemente acuitesi a causa delle conseguenze della crisi finanziaria ed economica internazionale e delle sue gravi ripercussioni all'interno dell'Unione europea. Le fibrillazioni che stanno investendo i principali Paesi europei sono, d'altra parte, sotto gli occhi di tutti. Tali imprescindibili esigenze di rigore hanno, inoltre, precluso al nostro Paese - così come, ad esempio, a Spagna e Svezia - di fornire proiezioni sul proprio impegno finanziario per il triennio 2011-2013,

per cercare di individuare le risorse da destinare al Fondo globale contro l'AIDS e definire i possibili contributi per il prossimo triennio. In quest'ultimo caso, ogni iniziativa legislativa richiede, come noto, l'indicazione di un'idonea copertura finanziaria, compito che appare al momento di non facile soluzione. Ciò nonostante, l'Italia, grazie anche all'attiva partecipazione costantemente mostrata nell'elaborazione delle strategie del Fondo e nei lavori dei suoi comitati e in virtù di un consistente impegno finanziario pregresso, mantiene un seggio nel consiglio di amministrazione (*Board*), formando un raggruppamento con la Spagna, effettivo dal gennaio scorso. Nel *Board* il raggruppamento italo-spagnolo occupa uno degli otto posti assegnati ai membri donatori. L'impegno italiano nella lotta alle grandi pandemie e, più in generale, nella cooperazione in campo socio-sanitario continua a rispondere sul piano bilaterale ad una precisa scelta di priorità settoriali della cooperazione allo sviluppo italiana, come indicato espressamente nelle linee strategiche della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri per il triennio 2011-2013. Circa l'iniziativa «*Education for all-Fast Track*», il nostro contributo complessivo nel 2011 è stato pari a 2,7 milioni di euro. Stiamo attualmente valutando l'entità del nostro futuro contributo in previsione della Conferenza dei donatori dell'EFT-FTI dell'EFT-FTI che avrà luogo a novembre. Infine, per quanto attiene a UN Women, il nostro Paese sta seguendo i primi passi dell'organismo nato nel 2010 e intende contribuire per sostenerne le importanti iniziative. Nel 2011 abbiamo fornito un contributo di 700.000 euro. Valuteremo, alla luce dei fondi che si renderanno disponibili in sede di legge di stabilità 2012-2014, la possibilità di contribuire ulteriormente alle attività di tale organismo.

Come ricordato dal senatore Di Giovan Paolo, la maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, includono i finanziamenti in favore della lotta ai cambiamenti climatici nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo Questa scelta può essere ricollegata a due principali ragioni. La prima è che l'ambiente rientra tra i principali settori in cui la cooperazione internazionale interviene per sostenere la crescita economica e il benessere dei Paesi in via di sviluppo, come previsto anche dagli obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite. La seconda ragione è che la tutela dell'ambiente è un obiettivo perseguito non solo attraverso programmi e progetti strettamente dedicati a tale ambito, ma anche mediante quelli focalizzati allo sviluppo di altri settori, come quello agricolo o quello idrico, collegati al rispetto ambientale. Come ricordato dall'onorevole interrogante, in occasione del Consiglio europeo del dicembre 2009 i capi di Stato e di Governo dell'Unione europea si sono impegnati a sostenere l'attività di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici da parte dei Paesi in via di sviluppo nel periodo 2010-2012 con 2,4 miliardi di euro all'anno, pari a 7,2 miliardi nel triennio. Si tratta dell'iniziativa definita "*Fast Start*". Tale impegno è stato riconfermato dall'Accordo di Copenaghen. Pur nella difficile congiuntura di finanza pubblica, il Governo italiano è da tempo impegnato, attraverso la Farnesina e il Ministero dell'ambiente, in un processo di inclusione delle questioni ambientali, e in particolare dei cambiamenti climatici, nelle strategie più generali di riduzione della povertà. Le linee guida della cooperazione italiana per il triennio 2011-2013 hanno infatti confermato le politiche ambientali, con particolare attenzione ai temi della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, tra i settori di intervento prioritario. In questo quadro, sono in fase di finalizzazione le linee guida ambiente, che recepiscono i principali orientamenti internazionali in materia di politica ambientale. In linea con gli impegni assunti a livello internazionale, la Farnesina contribuisce ai programmi di lotta ai cambiamenti climatici, inclusi quelli legati all'iniziativa europea "*Fast Start*", con stanziamenti pari a 460 milioni di euro per il triennio 2010-2012 (161,3 milioni per il 2010; 160,6 milioni per il 2011 e 137,6 milioni per il 2012). A queste cifre vanno aggiunti i 50 milioni di euro stanziati per il 2010 dal Ministero dell'ambiente. Il significativo incremento del contributo 2010 della cooperazione italiana a progetti ambientali, evidenziato dal senatore interrogante, è da ricollegare al fatto che, su richiesta dell'Unione europea e d'intesa con il Ministero dell'ambiente, si è provveduto nel 2010 ad effettuare una più ampia verifica che ha consentito di tracciare un quadro più completo ed esaustivo sull'effettivo impegno italiano nella lotta ai cambiamenti climatici. Per quanto riguarda le attività della cooperazione italiana, si rileva che la maggioranza degli interventi, realizzati prevalentemente in Medio Oriente, Africa e Asia, riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici con molteplici azioni dirette a ridurre la vulnerabilità dei sistemi umani e naturali agli effetti dei cambiamenti climatici, favorendo anche scelte di politica economica sostenibili da parte dei Paesi beneficiari. Le iniziative sono incentrate anche sull'uso di tecnologie pulite e su scelte di sviluppo economico a bassa intensità di carbonio e consistono altresì in interventi definiti "REDD+" (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*), attuati prevalentemente in Asia, Medio Oriente e America Latina, diretti ad affrontare il problema della deforestazione e della riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dalla deforestazione. Il principale canale di finanziamento è rappresentato dal credito d'aiuto, peraltro ad elevato tasso di iniziative di concessione (oltre il 70 per cento), a fronte del 30 per cento di iniziative finanziate a dono. Per quanto riguarda in particolare gli stanziamenti del Ministero dell'ambiente, che possono essere considerati come aiuti "a dono", va precisato che le risorse destinate a sostegno di misure di adattamento sono circa 14 milioni di euro, e quelle destinate a sostegno delle misure di mitigazione sono circa 31 milioni di euro. Inoltre, circa 4 milioni di euro sono stati destinati a misure volte alla riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione, misure che hanno effetti sia in termini di mitigazione sia in termini di adattamento, in linea con le indicazioni dell'Accordo di Copenaghen che invita le parti a destinare le risorse in maniera bilanciata (e non necessariamente uguale) e a dare priorità alle aree più vulnerabili. Si tratta di un approccio pienamente seguito dal Ministero dell'ambiente che ha attivato un'attività di cooperazione con gli Stati delle piccole isole del Pacifico. Per fornire un quadro dettagliato dei programmi attivati dalla Farnesina e dal Ministero dell'ambiente, sono lieta di consegnare ai servizi dell'Assemblea copia di un documento del Consiglio ECOFIN che riassume gli interventi italiani nell'ambito dell'iniziativa "*Fast Start*". Alla luce di queste azioni concrete, il Governo conferma quindi pienamente il proprio impegno a sostenere programmi e progetti a livello internazionale nel settore della protezione ambientale e dei cambiamenti climatici.

un sommario di riflessione su quella che dovrebbe essere una politica estera del Paese, che prescinde quindi dalle posizioni politiche, ma che, anzi, trae da queste le possibilità di soluzione. In primo luogo, non sono soddisfatto perché i dati

quell'occasione per cui qualsiasi argomento viene affrontato in un'Aula parlamentare viene scusato perché c'è la congiuntura economica (a parte il fatto che ritengo che proprio nella congiuntura economica si esalta il ruolo della politica, che dovrebbe disporre quando spendere e quando no: qui dovremmo fare più politica, e non meno). Detto questo, che è una mia opinione - spero condivisa da qualcuno altro - è evidente - ripeto - che dal 2008 abbiamo sospeso una serie di attività, ed è una scelta politica fatta anche mettendo in difficoltà parti attente e sensibili dell'attuale maggioranza rispetto a questo tema. Ho avuto modo in quest'Aula in altre occasioni di ringraziare il sottosegretario Mantica per il lavoro compiuto sulla cooperazione, ma non posso dimenticare che, appena eletti nel maggio del 2008, in un DPEF che ancora non teneva conto di alcuna congiuntura, la cooperazione allo sviluppo è stata ridotta già allora del 40 per cento, e sul 60 per cento che era rimasto c'è stata un'ulteriore riduzione l'anno dopo del 40

sviluppo è una funzione della nostra politica estera - quindi anche gli aiuti allo sviluppo dal punto di vista ambientale per l'importanza oggi della *green economy* sono parte della nostra politica estera noi tutti, a qualunque schieramento apparteniamo, dovremmo ritenere che, soprattutto nella congiuntura economica, non andrebbero fatti certi tagli. Avrà letto prima di me,

e di Gruppo, ma non ho alcun timore di dire che sono grato, una volta presa la decisione, a quelli che rappresentano il nostro Paese nelle Forze armate nonché ai cooperanti all'estero. Se però tagliamo sulle missioni, sulla nostra cooperazione, sulla cooperazione ambientale, sugli aiuti che diamo all'estero, sulla nostra presenza rispetto alle Nazioni Unite,

A livello internazionale, per la poca esperienza che ho riguardo ai temi europei, si mandano le proposte prima, e non si arriva all'ultimo momento: lo sappiamo, e noi abbiamo queste capacità. Allora, chiedo che da questa

il primo da esercitazione a corta gittata, con caratteristiche tecniche per un impiego esclusivamente addestrativo; il secondo «NATO Parabellum Standard», ordinariamente in dotazione al personale per i servizi di istituto. Le cartucce calibro 9x19 da esercitazione a corta gittata sono state acquistate dalla ditta Sellier & Bellot, avente sede nella Repubblica ceca, con procedura di aggiudicazione dell'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa, valutata da una commissione di gara, che si è avvalsa dell'attività di specialisti e di strutture dell'Esercito. In particolare, una prima fornitura di 10 milioni di cartucce è stata aggiudicata nel 2008 mediante procedura negoziata, ai sensi del codice dei contratti pubblici, dopo l'espletamento, con esito negativo, di una licitazione privata campionata. Ad entrambi i procedimenti di gara hanno partecipato sia la ditta citata Sellier & Bellot, sia la Fiocchi Spa. Una seconda fornitura di 6 milioni di cartucce è stata aggiudicata nel 2010 mediante gara europea con procedura ristretta, alla quale hanno partecipato le medesime ditte.

previo superamento delle prove previste da un capitolato tecnico - denominato STANAG NATO 4090 - adottato da tutti i Paesi membri della NATO. I relativi contratti sono stati stipulati nel 2007 e nel 2009, rispettivamente per 7.500.000 e 7.680.000 cartucce. La scelta di utilizzare, per quest'ultima fornitura, il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso è riconducibile all'esistenza, in tal caso, di un rigido capitolato tecnico, al quale i concorrenti dovevano tassativamente conformarsi. Per tutte le forniture, il collaudo è stato positivamente effettuato da un'apposita commissione. riguarda gli inconvenienti lamentati, accaduti durante l'attività di addestramento del personale della Polizia di Stato, sono state programmate le prove necessarie ad accertare se tali inconvenienti siano ascrivibili

Successive prove balistiche svolte in un poligono militare hanno evidenziato che le cartucce calibro 9x19 da esercitazione a corta gittata rientrano tutte nei parametri di prestazione previsti per questa tipologia di munizione. In seguito a tali verifiche tecniche, nello scorso mese di luglio è stata revocata la sospensione dell'utilizzo di circa 1.800.000 cartucce della stessa tipologia conservate nei magazzini di servizio degli uffici e reparti della Polizia di Stato. Per quanto riguarda, invece, le cartucce 9x19 NATO Parabellum, gli accertamenti finora disposti hanno mostrato che alcuni dei lotti acquistati non rientrano nei previsti parametri di sicurezza, e quindi non sono stati più utilizzati. l'attività di formazione e di addestramento de personale non ha subito interruzione. Infatti, le esigenze degli uffici a rischio di esaurimento delle scorte sono state soddisfatte mediante l'assegnazione di ulteriori aliquote di munizionamento, provenienti da future forniture. Per quando riguarda, poi, la giacenza attuale, quale scorta nazionale a disposizione per l'addestramento, la stessa è di circa 97.000 cartucce calibro 9x19 «NATO Parabellum Standard» e di circa 170.000 cartucce calibro 9x19 da esercitazione a corta gittata, oltre alle disponibilità di ciascun organismo della Polizia di Stato. Ricordo che nella programmazione ordinaria per l'anno 2011, tramite gara pubblica in ambito UE/WTO, è prevista la fornitura di complessivi 4.000.000 di cartucce 9x19 «NATO Parabellum Standard», di cui 800.000 prive di metalli pesanti negli inneschi e di vapori di piombo, nonché un ulteriore acquisto di 900.000 cartucce calibro 9x19 da esercitazione a corta gittata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

sottoscritto dal direttore logistico del Ministero dell'interno che, in via cautelativa, ha giustamente ritirato dall'utilizzo nella fase di addestramento i lotti del munizionamento difettoso. Intanto, prendo atto che il Governo ha confermato gli inconvenienti. Credo che in un Paese democratico non vi sia, anche su questioni che attengono la sicurezza interna e gli aspetti di tecnicalità che riguardano l'uso consentito

sua preziosa attività lavorativa non solamente quando è impegnato nelle situazioni di ordine pubblico, che sono visibili a tutti, ma anche quando è impegnato negli aspetti di preparazione e mantenimento della propria professionalità. Il dato di conferma e trasparenza che il Governo ha voluto indicare al Parlamento è un fatto apprezzabile.

una sorpresa - perché non era tema dell'interrogazione e non era nemmeno un dato conosciuto

dato risultati positivi. Come ha precisato il Sottosegretario, alcuni *stock* non rientravano negli standard richiesti dalla gara.

di possibile dialogo con il Governo su questi temi, una sanzione. Una rilevata inaffidabilità delle società che gestiscono forniture tanto importanti, non solo per la sicurezza dei cittadini, ma anche per la sicurezza dell'operatore di polizia,

nella legge n. 55 del 2002, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto a ciclo combinato della potenza di 385

del Ministero dello sviluppo economico è il prodotto di un procedimento molto complesso nel quale sono oggetto di un'attenta valutazione tecnico-amministrativa tutti gli aspetti territoriali e nel quale vengono presi in accurata considerazione i pareri di tutte le amministrazioni e degli enti coinvolti. In particolare, l'istruttoria si conclude una volta acquisiti la favorevole valutazione d'impatto ambientale sul progetto presentato, i pareri del Comune e della Provincia nel territorio in

a condizione che la società rispettasse una serie di condizioni e prescrizioni, tra cui l'esito negativo della procedura autorizzativa riguardante altra centrale da realizzarsi nella medesima macroarea. A valle del rilascio del decreto di VIA da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela in atto tutte le attività propedeutiche alla conclusione del procedimento tra cui, in particolare, quello per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Inoltre, al fine di pervenire alla conclusione dell'istruttoria, sono state svolte tre riunioni della Conferenza dei servizi, a carattere istruttorio, le cui risultanze sono contenute nei relativi resoconti Pertanto, considerato che in occasione della riunione del 16 dicembre 2009 non è stato possibile acquisire l'intesa regionale, causa l'assenza del rappresentante regionale, il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver approfondito ulteriori aspetti tecnici, ha dichiarato conclusa l'istruttoria comunicando che avrebbe convocato un'ulteriore riunione della Conferenza dei servizi. La giunta regionale della Campania, con nota del 20 ottobre 2010, ha trasmesso la deliberazione di Giunta regionale n. 691 dell'8 ottobre 2010 con cui ha espresso intesa favorevole all'autorizzazione in oggetto. Contro questa deliberazione il comune di Benevento ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della stessa nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente. Il tribunale del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione proposta dal Comune beneventano.

del 10 novembre 2010, il Ministero dell'ambiente ha comunicato il venir meno di questa condizione. Con nota del 12 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto a comunicare a tutte le amministrazioni ed enti facenti parte della conferenza dei servizi che, alla luce dell'intesa regionale, nonché della nota del Ministero dell'ambiente non si è ritenuto necessario procedere alla convocazione di un'ulteriore riunione della Conferenza dei servizi. Tali osservazioni sono state avanzate dalla Provincia di Benevento congiuntamente al Comune di Benevento, nonché dall'associazione "Altrabenevento", soggetti ai quali il Ministero ha fornito riscontro con separate note del 21 dicembre 2010. il nostro Ministero, a seguito di approfondimenti interni, con nota del 10 dicembre 2010, ha ritenuto opportuno richiedere l'avviso della commissione VIA circa la validità del giudizio favorevole già espresso con decreto del Ministero dell'ambiente, nonché circa il permanere della condizione che subordina il il giudizio favorevole espresso per la centrale in oggetto all'esito negativo della procedura autorizzativa, afferente altra centrale termoelettrica. La commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale ha confermato la validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso col citato decreto del 1° agosto 2008 ed ha ritenuto che fosse venuta meno la condizione indicata al punto n. 1 del quadro prescrittivo del succitato decreto di compatibilità ambientale, sulla base delle mutate condizioni di fattibilità previste inizialmente dalla delibera di giunta regionale n. 3533 del 2003, sostituita dalle disposizioni contenute nel piano energetico ambientale regionale. Pertanto il Ministero, sulla base degli atti sopra descritti, ha provveduto ad emanare il decreto 55/04/2010 del 21 dicembre 2010, con cui si autorizza la società Luminosa alla realizzazione dell'impianto in oggetto. Il 19 febbraio scorso, la società Luminosa ha pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto di autorizzazione, unitamente ad un estratto della VIA e l'8 marzo ha dato notizia dell'avvenuta emanazione del medesimo decreto su un quotidiano. Si rileva, infine, che il procedimento, condotto ai sensi della legge n. 55 del 2002, è avviato su istanza di parte e che il Ministero è tenuto al rilascio dell'autorizzazione unica a seguito di pronuncia di compatibilità ambientale favorevole e di favorevole intesa della Regione interessata, una volta conclusa positivamente l'istruttoria di competenza. Per quanto concerne le determinazioni assunte dalla Regione Campania con la soprarichiamata delibera, esse attengono all'autonomia dell'ente regionale in materia energetica. Si precisa che il consorzio ASI ha archiviato il procedimento di revoca del lotto assegnato alla società Luminosa, in quanto sulle medesime particelle è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio. Si rappresenta inoltre che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si svolge presso il Ministero dell'ambiente e, in tale ambito, ricade la circostanza evidenziata dall'interrogante circa un'istruttoria supplementare. Al riguardo, si informa che lo scorso 1° febbraio si è svolta la seconda riunione della conferenza di servizi, che si è conclusa con esito favorevole, in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica in oggetto. Si evidenzia, infine, che la sentenza della sezione sesta del Consiglio di Stato del 1° luglio 2008 ha sancito l'inesistenza di qualsiasi nesso teleologico e legame di presupposizione tra autorizzazione integrata ambientale ed autorizzazione unica,

e anche per comodità, non è stato precisato come il Ministero dell'ambiente abbia comunicato che è venuta meno la condizione di mancata realizzazione di un'altra centrale elettrica

riservandomi comunque di riprodurre altra interrogazione, signor Sottosegretario) che la Regione Campania ha espresso nella sua autonomia - così come lei ha precisato - la propria intesa, ma mi mi lascia perplesso il fatto che il Ministero dell'ambiente non abbia provveduto a fare un'istruttoria suppletiva.

sono rappresentante. Certamente non ci lascia soddisfatti il fatto che il parere del Comune, della Provincia e degli enti territoriali che rappresentano i cittadini, oltre ad una quantità incredibile di associazioni, a cominciare dell'associazione "Altrabenevento", si oppongono in maniera ferma, determinata

a produrre alcunché per quanto riguarda il *deficit* energetico che affligge l'Italia, e specialmente la nostra Regione Campania.

Ringrazio la Presidenza ed il Sottosegretario, ma mi devo lamentare soprattutto con il Governo, in quanto non è possibile rispondere ad un'interpellanza dopo 14 mesi: resto veramente sconcertato. Io credo che un Governo debba anche rispettare la rappresentanza che noi abbiamo del nostro territorio. Noi crediamo nelle nostre comunità; non vogliamo chiuderci in noi stessi, ma vogliamo rappresentare anche le difficoltà delle nostre comunità, e un Governo che tiene al Paese penso che debba assolutamente darci retta.

che dimostrò l'impotenza della scienza, l'impotenza umana, che durò tanti e tanti mesi, per tamponare una falla di petrolio, con l'inquinamento di un intero golfo e di diverse regioni dell'America Centrale e dell'America del Nord. Contemporaneamente, signor Sottosegretario,

Non si è seguito neanche il consiglio dello stesso presidente Obama che, dopo quel famoso disastro, ha invitato tutti ad un momento di riflessione. porterei lontano il discorso, anche sul tipo di sviluppo economico che noi dobbiamo assolutamente portare avanti, anche perché - vado subito al sodo, signor Sottosegretario - innanzitutto vanno fatte delle scelte

Zingaretti ed altri si sono mossi per poter salvaguardare quel lembo di terra. Ne approfitto, signor Sottosegretario, per dire al Governo che bisogna fare questa scelta e bisogna dire no

di alcuni pozzi di estrazione di antica data. Credo spetti anche al Molise avere determinate *royalty* per il proprio sviluppo locale.

Vogliamo innanzitutto precisare - questo la dice lunga su alcuni fenomeni che, anche da un punto di vista comunicativo, con il massimo rispetto, ritengo siano a volte frutto dell'immaginazione che, a seguito delle nuove norme di protezione ambientale particolarmente restrittive, introdotte dal decreto legislativo n. 128 del 2010, non è stato autorizzato nessun nuovo sondaggio, né l'esercizio di alcuna nuova piattaforma mobile di perforazione mentre, al contrario, sono state rigettate 20 istanze di richiesta di ricerca e fermati investimenti di ricerca per circa 190 milioni di euro. Le notizie riportate in merito dagli onorevoli interroganti e riferite come da fonti qualificate si confermano quindi destituite da ogni fondamento. Premesso ciò, in riferimento alle procedure di valutazione dei rischi legati all'attività estrattiva, si fa presente che queste sono state condotte con il massimo rigore scientifico, sulla base del principio di precauzione. Si ribadisce che la costa del medio-alto Adriatico è soggetta a rilevazione altimetrica e i relativi dati sono regolarmente trasmessi alle Regioni interessate. Sono inoltre attuati i protocolli di rilevazione della subsidenza - fenomeno consistente nel lento e progressivo abbassamento verticale del fondo di un bacino marino o di un'area continentale - prescritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio I sistemi di sicurezza degli impianti estrattivi *offshore* sono stati analizzati e verificati e sono stati approntati adeguati piani di emergenza. In particolare, i piani di protezione e le tecniche utilizzate per l'estrazione degli idrocarburi sono descritti dettagliatamente nei documenti di sicurezza e salute, disposti dalle società ENI ed Edison e depositati presso l'autorità di vigilanza. Inoltre, le conseguenze di un possibile incidente, legato all'attività estrattiva *offshore* in Adriatico, sono state ampiamente analizzate e valutate. Il Governo italiano ha attivato una campagna di controlli straordinari su tutti i pozzi petroliferi in mare, con esito positivo, ed ha costituito un gruppo di esperti nell'ambito della commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie al fine di valutare le cause e le circostanze dell'incidente del Golfo, ed i cui lavori conclusivi sono stati presentati a luglio dello scorso anno. Il gruppo di lavoro della commissione ha concluso le proprie attività sulla base dell'esame delle procedure di sicurezza nelle operazioni e dei piani di emergenza in caso di incidente, considerando gli esiti dei confronti con gli operatori (ENI, Shell ed Edison). Si fa presente, poi, che i titolari delle attività di ricerca e di coltivazione di idrocarburi sono responsabili degli eventuali danni ambientali prodotti e sono sottoposti dalla legge a obbligo di ripristino. Dopo l'incidente nel Golfo del Messico l'Unione europea si è impegnata sullo sviluppo, con il contributo italiano, di nuove direttive che prevedono anche strumenti assicurativi e di garanzia per eventuali grandi incidenti *offshore*. Nell'ambito del protocollo *offshore* della Convenzione di Barcellona, che l'Italia sta ratificando, è prevista l'adozione di norme e di procedure appropriate per stabilire le responsabilità ed i risarcimenti per i danni derivanti dalle attività. Il protocollo impegna le parti contraenti a prevedere che gli operatori siano responsabili per i danni causati dalle attività e che siano obbligati a pagare prontamente e con adeguati indennizzi. Sarà pertanto prevista l'adozione di tutte le misure necessarie per garantire che gli operatori abbiano una copertura assicurativa o altra garanzia finanziaria. Con i recenti decreti ministeriali 4 e 22 marzo 2011, il Ministero ha stabilito le procedure operative per lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

L'articolo 28 del decreto legislativo n. 128 del 2010 sopra citato, dal canto suo, prevede che, qualora dall'esecuzione dei lavori, ovvero dall'esercizio dell'attività derivino gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente possa ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare. Infine, si fa presente che il comparto per la ricerca e l'estrazione petrolifera in Italia occupa 65.000 addetti, compreso l'indotto, e produce entrate fiscali e *royalty* per oltre un miliardo di euro l'anno. Dal punto di vista dell'incidenza di rischi per l'ambiente, si osserva che nei 50 anni di storia produttiva trascorsi nell'Adriatico, non si sono verificati incidenti o inquinamenti di sorta. Si tratta di dati facilmente desumibili dal fatto che la pressione e la profondità alle quali si trovano i giacimenti ancora in attività nel mare Adriatico sono infinitamente inferiori a quelle

del fatto che certe autorizzazioni non devono essere concesse, nella maniera più assoluta. Bisogna fare delle scelte di ordine e di sviluppo o da un punto di vista turistico o da un punto di vista economico. Sentivo parlare prima della centrale a turbogas, e chiaramente

giustamente in positivo sotto tanti aspetti, dobbiamo parlare di federalismo anche nella produzione di energia elettrica e di altro, che pesa sull'ambiente di alcune nostre comunità.

il Governo renderà un'informativa sull'incidente avvenuto in una fabbrica di Arpino, nonché sulla crisi dello stabilimento Irisbus di Valle Ufita, in provincia di Avellino. I rappresentanti dei Gruppi potranno intervenire per cinque minuti per ciascuna informativa.